non era stato presentato in maniera pubblica e quindi non era dato conoscere i dati ufficiali. Noi eravamo ancora in presenza soltanto di un comunicato del maggio 2005 e sul sito ufficiale delle Ferrovie questi dati di bilancio non venivano presentati. Avevamo poi delle informazioni sommarie rispetto alla semestrale, che si stava chiudendo con una perdita di 1.022

Questa è veramente un'anomalia, perché una società che è in perdita dovrebbe fare in modo di comprimere i costi, cercare di ridurre gli sprechi e fare quelle operazioni perlomeno di

al Ministro dell'economia e delle finanze se era tollerabile che questo genere di aiuti da parte di una società pubblica in stato di gravissime perdite

la situazione economico-finanziaria del 1992. Chiedevo inoltre se non riteneva opportuno assumere per quanto di competenza iniziative concrete e urgenti al fine di evitare che società in perdita potessero sovvenzionare surrettiziamente della fiscalità generale manifestazioni che dovrebbero essere invece unicamente finanziate dai soci, oppure dalle comunità locali, dai governi locali, rispetto ai quali questi soggetti fanno riferimento.

966, 967, 968 e 969 (proprio quelli che fanno riferimento al gruppo Ferrovie dello Stato), medesima. Questa anomalia «illuminava» la vicenda del bilancio delle Ferrovie nella sua interezza, perché tali commi servivano a costruire il bilancio del gruppo Ferrovie dello Stato.

e dopo l'approvazione della legge finanziaria) e se non si riteneva conforme alla normativa vigente sulle società per azioni che il bilancio 2005 della *holding* gruppo Ferrovie dello Stato non

situazioni ormai intollerabili. Per queste ragioni, mi attendo dal rappresentante del Governo, che ringrazio

Vi fu poi una serie di contatti con i rappresentanti della fondazione al fine di verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per la definizione di un accordo, al quale Trenitalia decise infine di aderire. L'accordo fu siglato il 10 luglio 2006. Il «Romaeuropa Festival» rappresenta, nel proprio settore, una delle più rilevanti manifestazioni europee e pertanto è stata considerata l'opportunità di diffondere tra le diverse migliaia di partecipanti agli appuntamenti del Festival la conoscenza delle nuove *fidelity card* di Trenitalia destinate alla clientela (ovvero le quattro Carte Viaggio che avevano sostituito le precedenti Intercity Card e Carta Club Eurostar). La partecipazione alla sponsorizzazione del «Romaeuropa Festival» è stata ritenuta, quindi, un valido canale per la diffusione di nuovi prodotti, oltre che di acquisizione di clientela e di promozione, avendo, peraltro, Trenitalia, in qualità di *main sponsor*, la possibilità di accedere ad una serie di iniziative collegate alla manifestazione, particolarmente efficaci sotto l'aspetto della comunicazione e del *marketing*. Per quanto concerne le condizioni economiche, la società Ferrovie dello Stato ha precisato che l'accordo raggiunto con la Fondazione Romaeuropa - a fronte di un importo complessivo contrattualmente determinato in 54.500 euro più IVA ha comportato per Trenitalia un esborso effettivo, al netto dell'IVA, di 29.500 euro (in quanto la parte restante è stata, di fatto, compensata dall'acquisto, da parte dell'organizzazione, di spazi sui canali di diffusione e comunicazione di Trenitalia), quindi, ad un quinto il proprio impegno economico, rispetto alla cifra inizialmente richiesta dall'organizzazione e mantenendo, comunque, le medesime caratteristiche di partecipazione (ovvero ruolo di *main sponsor* e prerogative connesse). L'impegno finanziario di Trenitalia per la sponsorizzazione in questione riguarda peraltro l'esercizio 2006; attualmente, in considerazione della situazione economica contingente, sono sospese tutte le attività del medesimo genere che implichino impegni economici di qualsiasi importo.

Del resto, ne fa conferma il fatto stesso che l'intervento della finanziaria sia giunto proprio per determinare le nuove condizioni di bilancio.

all'estero - la Rete ferroviaria italiana ha fatto una grande campagna pubblicitaria per quanto attiene alla rete.

potrei affermare che l'analisi del bilancio 2005 induce a molte valutazioni e considerazioni a fronte delle riduzioni del valore della produzione.

Presidente, le Ferrovie dello Stato ci hanno comunicato quanto segue. La linea Torino-Ivrea è servita sia da collegamenti diretti con tempi di percorrenza di circa 50 minuti, che da treni regionali inseriti nell'intervallo di quelli diretti, tutti in cadenzamento orario. I monitoraggi effettuati nei primi tre mesi dell'anno in corso hanno rilevato che le *performance* di puntualità nella fascia di arrivo entro 5 minuti dall'orario previsto, hanno avuto un graduale miglioramento rispetto all'analogo periodo del 2006. In particolare, nei mesi di gennaio e febbraio 2007, gli *standard* di puntualità entro la fascia 0-5 minuti hanno superato l'86 per cento, mentre quelli nella fascia 0-15 minuti, il 98 Per quanto attiene ai treni in servizio, al fine di migliorare la qualità e il *comfort* di viaggio per i passeggeri, Trenitalia, in accordo con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ha definito un programma finalizzato al rinnovamento dell'attuale parco rotabile, prevedendo l'acquisizione di nuovi treni. In particolare, a seguito dell'accordo con la Regione Valle d'Aosta, a partire dal mese di giugno 2007, sulla linea Torino-Ivrea-Aosta saranno immessi in circolazione 9 treni «Minuetto» di ultima generazione. Inoltre, sul collegamento Chivasso-Ivrea, a seguito del completamento dei lavori di elettrificazione della linea, verrà impiegato anche materiale elettrico più recente rispetto a quello *diesel* attualmente in circolazione. Peraltro, il recente incremento degli interventi di manutenzione, effettuati sul materiale rotabile nei primi mesi del 2007, ha comportato una sensibile diminuzione del ricorso alla soppressione dei collegamenti per guasti, riduzione quantificabile intorno al 60 Per quanto concerne la sicurezza a bordo del treno, oltre all'intensificazione dei controlli, tesi a limitare il fenomeno dell'evasione dei biglietti ferroviari ed a migliorare l'assistenza alla clientela, sono state poste in essere le seguenti iniziative finalizzate a tutelare maggiormente la sicurezza dei passeggeri: passeggeri: agevolazioni tariffarie per i funzionari delle forze dell'ordine che forniscono assistenza al personale di scorta treni; servizio di assistenza alle fasce deboli (anziani, scolaresche, eccetera) svolto su alcuni treni da parte di agenti di polizia a riposo dell'ANPS (Associazione nazionale Polizia di Stato); infine, installazione di sistemi di videosorveglianza a bordo per il materiale rotabile rinnovato (il nuovo materiale è già dotato di tale dispositivo). Per quanto riguarda la linea Torino-Milano, anche i monitoraggi effettuati sulla linea stessa nei mesi di gennaio e febbraio 2007 hanno rilevato un graduale e sensibile miglioramento delle *performance* di puntualità rispetto a quelle del medesimo periodo dell'anno precedente. Infatti, gli *standard* di puntualità nella fascia di arrivo entro i 5 minuti hanno superato il 91 per cento, mentre quelli della fascia 0-15 minuti si sono attestati intorno al 97 La società Ferrovie dello Stato ha precisato che le tariffe degli abbonamenti regionali del Piemonte attualmente in vigore sono ancora quelle adottate dal mese di ottobre 2002 e che da tale data non sono state oggetto di alcun aumento. Per quanto concerne, invece, gli aumenti tariffari dei collegamenti della media/lunga percorrenza attuati dal 1° gennaio 2007, questi consentiranno un recupero solo parziale del tasso di inflazione, permettendo, comunque, di avviare un progressivo riallineamento dei prezzi a quelli praticati dalle principali reti europee.

Credo, Presidente, che, se vogliamo ripristinare un corretto rapporto tra Parlamento e Governo, il Governo debba rispondere sotto la propria responsabilità e non possa venire qui a riferirci che cosa gli trasmettono le Ferrovie dello Stato, cioè una risposta assolutamente burocratica, senza alcuna valutazione critica rispetto a quanto viene indicato. Questo è il primo punto se vogliamo riprendere un dialogo forte tra Governo e Parlamento. Sono insoddisfatto, Presidente, per

Questi ritardi sono dovuti a guasti del materiale e delle strutture fisse, in modo particolare dei passaggi a livello, al tranciamento dei cavi dell'elettrificazione;

a tutt'oggi a senso alternato e a tratti ancora dotata di strutture provvisorie e precarie, si registrano fortissimi disagi e ritardi che sono stati parzialmente affrontati da Trenitalia con la soppressione della fermata di tutti i convogli, eccetto due, nella stazione di Settimo Torinese che - si ricorda - annovera l'utilizzo della linea da parte di migliaia di passeggeri al giorno e costituisce un nodo ferroviario importante per il collegamento con l'Alto Canavese tramite una ferrovia in concessione. La tratta Chieri-Settimo, gestita dal Gruppo Torinese Trasporti SpA, annovera problematiche sulla tratta Chieri-Torino Lingotto e in tali stazioni i convogli della società concessionaria devono concedere precedenza ai treni della società Trenitalia. A causa di ciò, nella percorrenza dei 18 chilometri che collegano Torino Lingotto-Settimo Torinese non infrequentemente si collezionano ritardi di oltre trenta minuti. Su tutti i treni si registrano sporcizia, mancanza d'acqua, di sapone e carta nei bagni; una carrozza su due chiusa a chiave; impianti di riscaldamento e condizionamento spesso non funzionanti; carenza di illuminazione; totale mancanza di controllo da parte del personale di bordo; porte non funzionanti nelle ore di punta o sovraffollamento. Problematiche poi si registrano ancora nelle stazioni a causa di eventi atmosferici. Le stazioni e Settimo Torinese sono vere e proprie piscine dove l'acqua gronda lungo le pareti degli impianti elettrici e sempre a Settimo da circa un anno una delle porte della biglietteria è chiusa. Questi sono i problemi dei pendolari di tutti giorni. Allora voglio dire al Sottosegretario

che devono trovare soluzioni forti. Presidente, vorrei leggere brevemente una lettera che ha scritto un lettore de "la Stampa" sul problema dei treni: «A Oulx scende dall'Intercity proveniente da Parigi un nutrito gruppo di ragazzi di età di media superiore evidentemente reduce da una vacanza in Francia. Salgo nello stesso vagone dove ho il posto prenotato per Torino e mi trovo nelle più squallide sporcizie: carte unte, fazzoletti sporchi, vasetti vuoti di yogurt e gelati, macchie ovunque. Sono persino schifata al pensiero di sedermi al posto assegnato. La mia domanda è questa: questi prossimi maturandi con abiti firmati, dotati di tutte le moderne tecnologie a partire dai cellulari all'ultimo grido, per caso sono anche forniti di genitori preposti alla loro educazione, oppure le regole del vivere civile sono diventate un *optional*?» Ecco,

dagli utenti, dagli utenti cittadini. Per queste ragioni, Presidente, sono insoddisfatto. Credo che molta strada debba essere compiuta se vogliamo realizzare il doppio obiettivo di bilanci sani e al tempo stesso un servizio efficiente e una cultura di rispetto della cosa pubblica che deve essere portata avanti con determinazione.

stata presentata il 27 giugno 2006. Infatti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2006 è stato autorizzato il pagamento delle somme dovute a titolo di compensazione finanziaria per l'anno 2003 ai Comuni beneficiari e alle Comunità montane interessate. Inoltre, con elenco del 7 giugno 2006, n. 476, a cura del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati trasmessi all'Ufficio centrale di bilancio n. 131 ordini di pagare, su apposito capitolo, le somme in argomento. In particolare, si precisa che l'ammontare del citato ristorno per i comuni delle province di Varese e Como è stato pari a circa 21.726.000 euro. Signor Presidente, ringrazio lei ed il Sottosegretario. So perfettamente che il Governo ha trovato una soluzione al problema che ho rappresentato nell'interrogazione e potrei dichiararmi parzialmente soddisfatto proprio per quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario. Tuttavia, c''è un piccolo aspetto che voglio ricordare,

Peraltro, so che su questi fondi frontalieri si gioca veramente la sopravvivenza di tanti piccoli Comuni delle nostre valli e dei nostri laghi, dal momento che sono purtroppo - purtroppo - o per fortuna, dipende dal punto di vista - un cittadino quasi della Svizzera meridionale, essendo stato eletto in Lombardia, ma risiedendo a Como. Molti dei nostri Comuni rivieraschi, del lago e delle valli, vivono grazie al ristorno dei fondi frontalieri. Non è possibile distribuire sul territorio fondi frontalieri con questo ritardo: nell'estate 2006 sono stati erogati i fondi del 2003, come giustamente lei ha ricordato. Occorre velocizzare i tempi, perché su questi ristorni, ripeto, le piccole amministrazioni fanno un grande affidamento per realizzare interventi di pubblica utilità nei territori in cui risiedono i frontalieri, quindi è un atto dovuto. Credo che abbiate piegato la resistenza degli enti locali con l'ultima legge finanziaria: li avete costretti a fare peripezie per rimanere a galla sotto il profilo economico-finanziario (non ultima evidentemente, la possibilità di aumentare l'ICI). Non esagerate. Non esagerate con i tempi di risposta alle interrogazioni,

e le finanze*. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato che in base all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, gli uffici dell'Agenzia possono svolgere la propria attività di controllo, tra l'altro, attraverso l'accesso - cito testualmente - «nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni». Pertanto, sono legittime le ricerche presso i locali e i beni aziendali. L'Agenzia delle entrate ha riferito che, comunque, da quanto rappresentato anche dagli organi di stampa, alla stessa non risulta che si sia verificato alcun caso in cui i funzionari dell'Agenzia medesima hanno maneggiato direttamente il denaro contante presente in cassa ed inoltre che dagli stessi organi di stampa è stato, invece, riconosciuto che i medesimi funzionari si sono comportati con gentilezza e correttezza. Per quanto riguarda le istruzioni operative fornite ai funzionari che svolgono l'attività di controllo, si fa presente che dal 1997 sono state pubblicate le metodologie di controllo, quali strumenti di ausilio all'attività di verifica nei confronti degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali. Sul sito *internet* dell'Agenzia è pubblicato il testo delle metodologie di controllo delle piccole e medie imprese e dei professionisti. In tali metodologie viene indicato, tra le operazioni da seguire, il controllo della cassa al fine di verificare se i valori rinvenuti (siano essi denaro, ricevute di carte di credito e bancomat) trovano riscontro con gli incassi complessivi e parziali registrati al fine di individuare le modalità d'incasso. È altresì indicato che una certa differenza può essere giustificata da esigenze di funzionamento della cassa che richiedono una giacenza minima (per dare il "resto" o per esigenze improvvise). In particolare, la presenza in cassa di valori superiori al totale degli importi registrati va valutato quale possibile elemento indiziario sintomatico dell'esistenza di operazioni commerciali non contabilizzate. Quindi, la presenza di una differenza, tra le somme in cassa e quanto risultante dal totale degli scontrini, non riconnette automaticamente, quale unica motivazione, la mancata registrazione e quindi evasione di incassi, fiscalmente rilevanti. Comunque, all'interno di tipi di controllo più ristretti e mirati, come la verifica del rispetto degli obblighi strumentali relativi ai registratori di cassa, le risultanze dello specifico controllo in argomento, seppur con le cautele sopra evidenziate, devono essere tenute nella giusta considerazione. Per completezza di trattazione, si fa presente altresì che i controlli sul rispetto degli obblighi strumentali, tra cui il controllo sulle violazioni in materia di scontrino fiscale, rientra tra le attività tipiche, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate svolgono in attuazione della convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima con riferimento, in particolare, alla convenzione del 7 aprile 2006, in coerenza con gli indirizzi pluriennali contenuti nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia.

È evidente che ho per primo apprezzato la serietà ed il garbo con cui hanno inteso operare i funzionari dell'Agenzia delle entrate. Sta di fatto che la questione politica è ben più importante. Questo è solamente un piccolo fatto, perché il Governo si è abbattuto su commercianti ed artigiani come un tornado caraibico. In ordine all'evasione fiscale, per quanto concerne commercianti ed artigiani, il vice ministro Visco applica più che altro la presunzione di colpevolezza, non di innocenza, per cui secondo me, comunque, sei colpevole; dimostrami il contrario! Questa è la *ratio* di molti interventi del Vice ministro e, lo dico con un po' d'ironia, mi ha fatto pensare che i colleghi delle minoranze linguistiche, in particolare quelli eletti nell'Alto Adige, lo chiamano «fice ministro Fisco!». Questo è sintomatico anche dell'apprezzamento nei confronti del vice ministro Visco. Siamo tutti contro l'evasione fiscale, non ci sono i primi della classe, onorevole Sottosegretario. Ma c'è modo e modo per combatterla e, nel caso di specie, pensare che un commerciante, magari ambulante, lasci grandi somme nelle casse anziché metterle al sicuro da qualche parte, considerata la pletora di malintenzionati che circolano per i nostri mercati, è francamente fuori da ogni regola del buonsenso. Il controllo è giusto, ma l'oppressione è sempre molto fastidiosa.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano è venuta a conoscenza dell'intenzione del Comune di Blevio di intervenire sul complesso vincolato in seguito a diverse segnalazioni. Nel giugno 2006 la Soprintendenza ha inviato all'amministrazione comunale un primo parere negativo sull'entità e sulla qualità dell'intervento proposto per il complesso vincolato, ribadito successivamente nel settembre 2006, data l'assoluta incompatibilità delle opere in progetto con lo stato dei luoghi. Essa ha inoltre ritenuto di richiamare il Comune al rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, evocando gli estremi del provvedimento di vincolo diretto sull'intero complesso e ricordando altresì la necessità di sottoporre al suo esame qualsiasi intervento di modifica del bene ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004. II complesso di Villa Rocca Bruna risulta invece sottoposto a vincolo paesaggistico (decreto ministeriale 15 aprile 1958). II complesso è rimasto inutilizzato per circa vent'anni, fino a quando la nuova proprietà, d'accordo con il Comune di Blevio, ha deciso di realizzare una struttura alberghiera. II relativo progetto è stato autorizzato dal Comune che, in seno alla Commissione edilizia, ha espresso attraverso i suoi esperti ambientali un parere paesaggistico favorevole. La Soprintendenza invece ha annullato, per motivi di legittimità, quattro autorizzazioni sindacali nel 2003, nonché una nel 2004 ed ha espresso due pareri negativi in sede di Conferenza dei servizi nel 2006 in merito alla proposta di costruzione di una piscina galleggiante situata davanti alla Villa. È il caso di sottolineare che il Comune, nonostante i provvedimenti della Soprintendenza, ha più volte autorizzato il progetto sulla base di piccole ed irrilevanti modifiche. Occorre segnalare, inoltre, che il potere di controllo esercitato dalle Soprintendenze è limitato al mero esame dell'*iter* logico e motivazionale che ha portato il soggetto proposto alla gestione del vincolo ad autorizzare l'intervento. Da ultimo si evidenzia che la Regione Lombardia, con legge regionale n. 12 del 2005, ha sub-delegato la competenza in tema di tutela paesaggistica agli enti locali, in particolare ai Comuni, senza conservare alcun potere residuo. Pertanto, la responsabilità degli interventi assentiti sul territorio ricade sull'amministrazione comunale quale soggetto *in primis* competente alla gestione del vincolo. facoltà. BUTTI *(AN)*. Onorevole Sottosegretario, nulla di personale, anzi se crede, visto che anche le prossime interrogazioni sono sempre a mia firma, possiamo concludere alla *buvette* bevendoci un un caffè. Le esprimo tutta la mia solidarietà, perché lei è Sottosegretario alle finanze e viene a rispondere in ordine a temi per i quali probabilmente non ha alcun interesse e che non la affascinano. La risposta che lei ha garbatamente dato a quest'interrogazione, però, è preoccupante; non ho dubbi che il sindaco del Comune di Blevio sia un gentiluomo e un amministratore scrupoloso, non ho nemmeno dubbi che la sua amministrazione abbia seguito una procedura corretta, ma sono ugualmente preoccupato - e lo sono ancor di più alla luce di quanto ho sentito poc'anzi perché vivo, come dicevo prima, in un posto che ritengo incantevole, e credo che il lago di Como offra spettacoli incomparabili sotto il profilo delle bellezze artistiche, architettoniche, naturali, paesaggistiche; tanti piccoli Comuni di raro fascino si affacciano sulle sponde del Lario e non oso pensare cosa accadrebbe se tutti i sindaci e tutte le piccole amministrazioni cominciassero autonomamente e - per carità, come lei stesso ha riconosciuto, legittimamente - a promuovere progetti edilizi di un certo impatto visivo e non solo visivo. Giustamente lei ha ricordato che il potere di controllo della Soprintendenza è limitato, che la Regione non ha alcun potere di intervento e che la tutela paesaggistica è delegata per intero ai Comuni e questo può essere, come le dicevo, fonte di preoccupazione perché esattamente di fronte a Blevio, e quindi sulla sponda occidentale del Lario, un altro sindaco ipotizza passerelle a lago e funicolari futuristiche. Qualche altro sindaco, attirato dagli oneri di urbanizzazione o da altre entrate con cui sollevare le sorti economiche del paese amministrato e, ripeto, messo in ginocchio dalla finanziaria del vostro Governo, strizza l'occhio ai grandi gruppi interessati a realizzare opere certamente importanti ma altrettanto imponenti sulle sponde del lago. Sicuramente, molti di questi interventi saranno anche utili all'economia del turismo tradizionale e d'affari, ma ammetto che mi allarma che lei oggi ha ribadito, di un controllo del territorio efficace, efficiente e anche tempestivo che abbia una visione d'insieme del lago, del suo paesaggio e quindi del territorio, senza considerare solo

in futuro un disegno di legge che focalizzi l'attenzione delle autorità competenti su quello che è un problema importantissimo della gestione del territorio.

Come già riferito in sede di risposta alle precedenti interrogazioni riguardanti l'autorizzazione all'apertura della multisala Camerlata 2000, il Ministero per i beni e le attività culturali ha disposto accertamenti ispettivi sull'area interessata. L'ispettore incaricato ha affermato che sull'area in questione non è stata rilasciata alcuna autorizzazione avente ad oggetto l'apertura di un centro commerciale. È stato quindi chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla sussistenza - nella fattispecie del presupposto dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento o alla revoca dell'originario atto autorizzatore. L'Avvocatura generale dello Stato ha puntualizzato che l'interesse pubblico che potrebbe portare alla revoca del provvedimento autorizzatorio è riconducibile alla sfera di interessi di competenza delle amministrazioni locali. La direzione generale per il cinema ha quindi contattato il Comune di Como e la Regione Lombardia al fine di valutare la sussistenza o meno di un interesse pubblico attuale alla revoca del provvedimento amministrativo con il quale è stata autorizzata l'apertura della multisala Camerlata 2000. La Regione Lombardia, in data 22 dicembre 2006, ha comunicato di non avere competenza a riscontrare l'esistenza o meno di un interesse pubblico alla revoca del provvedimento. Il 20 marzo ultimo scorso il sindaco del Comune di Como ha comunicato che: «Dal combinato disposto dell'articolo 3, del decreto ministeriale n. 391 del 1998 e dell'articolo 4, comma 1, lettera *g),* del decreto legislativo n. 114 del 1998 emerge che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga, è previsto il riscontro di soli requisiti tecnico-oggettivi-fattuali. Ciò nel presupposto che il legislatore stesso ha già apprezzato, in precedenza e in astratto, l'interesse pubblico (qui evidentemente riferito a quello della libertà di intrapresa ed ai suoi riflessi socio-economici) sussistente ogniqualvolta risultino verificati quei requisiti di cui in precedenza, senza che i medesimi siano da riscontrarsi di volta in volta. Pertanto e conclusivamente, alla luce di quanto sopra, non pare che tale interesse pubblico possa considerarsi essere venuto meno, sussistendo all'attualità quei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.» II Comune di Como II Comune di Como ha altresì precisato che il piano territoriale della Provincia di Como è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 188 del 20 settembre 2006 ed ha acquistato efficacia solo dopo la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11 settembre 2006 dì adozione del cosiddetto PIR (Programma Quanto all'operato di questo Ministero, si rileva che l'istruttoria effettuata dalla direzione generale per il cinema è stata tutt'altro che carente, come si evince dal verbale della vista ispettiva e come è stato riconosciuto dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha espressamente affermato che «l'operato dell'amministrazione nella fase procedimentale che ha preceduto l'emanazione dell'atto di autorizzazione appare del tutto esente da censure.» Si sottolinea inoltre, che la citata segnalazione del 15 settembre 2000, oltre a riferirsi all'istruttoria di una precedente richiesta di autorizzazione - poi revocata per decorrenza dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori è stata seguita da altra nota del 21 settembre 2000 che descriveva la situazione come corrispondente alle prescrizioni normative e che anche allora, sottoposta all'esame della Commissione apertura sale cinematografiche nella riunione del 19 ottobre 2000, ne ottenne il parere favorevole al rilascio di autorizzazione. In merito alla notizia della chiusura della multisala, la direzione generale per il cinema è in attesa di ricevere le necessarie informazioni al fine di poter valutare se ricorrano o meno i presupposti previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 391 del 1998 per la decadenza dell'autorizzazione.

perché non voglio abusare neanche della disponibilità del Sottosegretario. Desidero far notare, non è la prima interrogazione che presento in ordine al problema della cosiddetta ex Trevitex e che, in più di un'occasione, non si è presentato a rispondere il rappresentante del Ministero competente ma sono stati delegati, in un caso, il sottosegretario all'interno Lucidi, e, nell'altro, lei, A me sembra che in questa vicenda affiori un dialogo tra sordi, perché è del tutto evidente che vi siano irregolarità, che emergono prepotentemente confrontando i documenti prodotti dai privati, dall'amministrazione comunale e dal Governo. Governo. Mi domando, allora, quando il Governo - cioè l'amministrazione - deciderà di non prendersi più in giro e di non prendere più in giro non solo l'interrogante (che, peraltro, preannuncia l'ennesima interrogazione, perché su questa vicenda intende andare fino in fondo) ma anche i cittadini di un intero quartiere di una città, che chiedono chiarezza su un episodio veramente oscuro. Come le dicevo, ho presentato interrogazioni - mi si dia atto di questo - tutte estremamente circostanziate, con dovizia di particolari

Dunque, chiediamo chiarezza. In quel quartiere, periferico rispetto al centro della città, che ha tanti problemi anche di natura urbanistica e viabilistica, evidentemente - come spesso accade alle periferie delle città non doveva e non poteva sorgere un centro commerciale, tanto meno un cinema multisala. Un centro commerciale lì non poteva in origine sorgere perché il Consiglio comunale lo aveva escluso tassativamente,

Quando verificherete, con le indagini che avete intenzione di espletare, i motivi che hanno portato alla chiusura di quel cinema, questi vi appariranno evidentissimi:

è un fatto di mercato. Como è una piccola città di 85.000 abitanti e la sua provincia ne ha 55.000: vi sono troppe sale cinema, per cui è evidente che lì il mercato non avrebbe consentito lunga vita ad un cinema multisala. Ma, per i cosiddetti - voglio utilizzare questa espressione - «furbetti del quartierino», l'esistenza dell'uno giustificava quella dell'altro: da ciò è nata un'incredibile produzione di atti amministrativi imbarazzanti. So già quale delle due versioni offerte dal Comune di Como - che giustamente l'amministrazione ha interpellato - presenti i requisiti dell'attendibilità, della credibilità e della serietà: basta leggere le carte per capire che il settore commercio di quel Comune non solo ha sempre, diligentemente risposto ai quesiti, ma ha mantenuto una condotta assolutamente trasparente e lineare in questi anni. In altri termini, leggendo quanto firmato dal dottor Di Giulio, chiunque capirebbe i termini della vicenda. Lei pensi che tutto quell'intervento urbanistico non era nemmeno inserito - come ha, forse ingenuamente, affermato anche il sindaco nella relazione nel piano territoriale di coordinamento provinciale. Lei pensi che il Consiglio comunale ha adottato un PIR dove si cita una legge regionale ritenuta esaurita. Lei pensi che è in corso una sorta di azione di *mobbing* strisciante sul funzionario comunale che ha «osato» rispondere, come sempre ha fatto, al Ministero.

ha ritenuto non ammissibile sotto il profilo urbanistico la richiesta, presentata da un noto *brand* della grande distribuzione, finalizzata a trasformare l'ex fabbrica in un centro commerciale; è quello che sostengo da dieci anni. Lei pensi che il cinema multisala, come giustamente ha ricordato, ha chiuso i battenti dopo diciotto mesi di attività, perché anche un babbeo avrebbe previsto la mancanza di mercato per quella struttura così vicina ad altre esistenti. E chi si assume la responsabilità dei 25 dipendenti licenziati? Allora, concludendo, sono profondamente insoddisfatto anche da questa risposta; ripresenterò l'ennesima interrogazione. A questo punto chiederò anche di essere ascoltato dalla competente procura della Repubblica, perché se sono un pazzo visionario, se i ricorrenti sono pazzi visionari, se un funzionario del Comune di Como è un pazzo visionario, bisognerà conclamare la questione; bisognerà che tutti, compreso il sottoscritto, vengano

che il Governo raccoglie le informazioni dove ritiene più opportuno, nel caso specifico alle Ferrovie dello Stato, ma va anche da sé che il Governo risponde e si assume per questo la responsabilità per le proprie competenze.